*question time*), sulla vicenda di una bambina bielorussa ospite di una famiglia genovese. Ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, dopo l'eventuale intervento del Governo un senatore per ciascun Gruppo parlamentare può,

Questo è quanto prescrive il Regolamento. Chiedo al ministro della solidarietà sociale, onorevole Ferrero, se intende intervenire preliminarmente. FERRERO, *ministro Signor Presidente, cercherò di riassumere i termini generali e specifici della vicenda, come contributo all'apertura della discussione, per permettere di affrontare meglio la questione.

Da tale fenomeno, nel corso degli anni, è scaturita l'esigenza di trovare un punto di incontro tra le attività delle associazioni e i compiti regolatori delle istituzioni al fine di consentire uno sviluppo adeguato del fenomeno.

535. È questo l'organo che si occupa dei minori stranieri non accompagnati e di quelli accolti.

per l'ingresso ed il soggiorno in Italia di tali minori, valutando l'affidabilità del proponente, la validità dell'iniziativa, nonché l'affidabilità del referente estero. Passo ora allo sviluppo della questione più direttamente in oggetto. La bambina di cui stiamo discutendo in questi giorni è Maroz Viktoryia, nata in Bielorussia il 25 maggio 1996; ha fatto ingresso in Italia nell'ambito di un programma solidaristico di accoglienza temporanea presentato dall'Associazione Puer ed approvato dal Comitato per i minori stranieri. Durante il soggiorno in Italia, la famiglia ospitante ha segnalato alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova che la minore avrebbe subìto violenze fisiche, psichiche e sessuali nell'internato dove era ospitata in Bielorussia. Iltribunale per i minorenni di Genova, dopo aver disposto, il 16 agosto 2006, l'affidamento della minore al Comune di Cogoleto, ove risiede la famiglia ospitante, per il tempo occorrente ai necessari accertamenti sanitari, in data 6 settembre 2006 ha disposto il rientro in patria della bambina nell'ambito di un programma di riabilitazione da far seguire alla minore, sulla base dell'impegno assunto in tal senso dalle autorità bielorusse, che hanno acconsentito alla permanenza temporanea nel loro Paese di sanitari italiani e della famiglia ospitante. Alla data prevista per il rientro in patria della minore, l'8 settembre 2006, la famiglia ospitante non si è presentata all'aeroporto e qui ha avuto inizio la vicenda della scomparsa della bambina. In seguito al ritrovamento della bambina, da parte delle forze dell'ordine, il 29 settembre 2006, in applicazione della sentenza emessa in data 7 settembre 2006 dal tribunale per i minorenni di Genova, la bambina è partita con un volo dall'aeroporto di Genova diretto in Bielorussia, accompagnata anche dalle due dottoresse italiane, la neuropsichiatra infantile Antonietta Simi e la psicologa Laura Battaglia della ASL 3 di Genova, nominate dal tribunale per i minorenni di Genova per seguire la riabilitazione della bambina in Bielorussia. Si segnala che nella citata sentenza veniva richiesto al Ministero degli affari esteri e a quello delle politiche per la famiglia, nonché alla Commissione per le adozioni internazionali, di informare periodicamente il tribunale di Genova sulla prosecuzione del trattamento della minore e sull'adempimento delle norme della Convenzione Convenzione dell'Aia ai fini della sua tutela. Passiamo ora alla vicenda in Bielorussia. All'arrivo in Bielorussia la bambina è stata trasferita in un istituto diverso da quello di provenienza, nella località di Borissov. I due I due medici italiani, unitamente all'*équipe* di specialisti bielorussi, hanno seguito la bambina e impostato il programma di riabilitazione della minore, così come previsto dalla decisione del tribunale per i minorenni di Genova. I due medici italiani, nel corso del loro soggiorno, hanno mantenuto contatti con l'Ambasciatore italiano e sono ripartiti per l'Italia l'11 ottobre scorso, ritenendo conclusa la loro missione. In seguito hanno informato l'Ambasciatore italiano di aver provveduto a inoltrare al tribunale per i minorenni di Genova una relazione sul lavoro svolto. In particolare, hanno indicato che le condizioni della minore sono buone dal punto di vista psico-fisico, aggiungendo che la bambina ha bisogno di un periodo di tranquillità per riprendersi dal carico emotivo degli ultimi tempi e riambientarsi in Bielorussia. Al riguardo, il Comitato ha seguito con la massima attenzione il caso in questione sin dal suo nascere, offrendo la piena collaborazione all'autorità giudiziaria e cooperando fattivamente con le altre amministrazioni competenti, nonché con la rappresentanza diplomatica bielorussa e in costante contatto con l'associazione proponente il programma di accoglienza, al fine di giungere ad una soluzione della vicenda che fosse la più adeguata alla tutela dell'interesse della minore. Il Comitato, che da anni gestisce programmi solidaristici di accoglienza temporanea che coinvolgono annualmente circa 25.000 minori bielorussi, auspica che la vicenda, che rappresenta un caso drammatico, possa concludersi nel rispetto delle determinazioni assunte dalla competente autorità giudiziaria. La strada sin qui percorsa dal Comitato, finalizzata ad individuare norme certe e chiare che regolino il fenomeno, è determinata dalla convinzione che, in fenomeni così delicati, non basti la buona predisposizione dei soggetti coinvolti ma occorrano regole istituzionali precise, che, oltre a svolgere una funzione di supporto e controllo alle iniziative solidaristiche, promuovano un'assunzione di responsabilità da parte del mondo dell'associazionismo della società civile. Si tratta di un'esperienza ormai ventennale che esprime concretamente l'alto livello di cooperazione tra l'amministrazione, la società civile e il Governo bielorusso. Questi sono i princìpi e gli obiettivi che il Comitato, anche nell'immediato futuro, perseguirà nella gestione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, il tutto sempre nel superiore interesse dei minori, per la loro completa tutela sia sotto il profilo delle leggi e delle convenzioni internazionali, sia per il rispetto dei princìpi educativi e dello sviluppo psichico dei fanciulli. Nello specifico (utilizzando ancora un un minuto, e poi ovviamente risponderò alle domande specifiche), vorrei sottolineare che il Comitato sta lavorando alla predisposizione di linee guida per il prosieguo dell'attività e dell'ingresso in Italia dei minori accolti, verificando se è possibile definire elementi normativi che tentino di evitare situazioni come quelle in cui ci siamo trovati. Questo lavoro è tuttora in corso; quindi, sarà mia cura dare informazioni, oltre che accogliere gli eventuali suggerimenti che potranno emergere dalla discussione di oggi, una volta che il Comitato, che riunisce vari Ministeri e varie amministrazioni e rappresentanze delle famiglie, abbia definito le linee guida su cui muoversi per il futuro.

i Gruppi regolano gli interventi: è prevista la possibilità di intervento per un senatore per ciascuno Gruppo parlamentare. parlamentare. Derogare a questa formula, anche organizzativa, significherebbe che un dibattito di questo tipo supererebbe

ad intervenire in questo dibattito. Le chiedo scusa se non posso farla intervenire. Ovviamente, la Presidenza sa quanto ella è sensibile a questo problema.

Le associazioni per i bambini di Chernobyl sostengono che, secondo uno studio dell'ENEA, un mese di ospitalità in Italia con un'alimentazione priva di radionuclidi permette a questi bambini Con due o al massimo tre di questi soggiorni si dovrebbe sanare un bambino. Perché, dunque, alcuni parenti dello stesso Lorenzetti ospitano lo stesso bambino da dieci anni? Perché la durata

anche qui ora, tra soggiorni terapeutici, adozione, affidamento ed affidamento internazionale. Affrontando il caso di una bambina abbandonata e strattonata da adulti

un controllo effettivo del Comitato per i minori stranieri, che afferisce al suo Ministero, sulle associazioni che si occupano di questi soggiorni estivi? Chi sceglie le famiglie italiane di accoglienza?

una volta conosciuto un bambino o una bambina di loro gradimento, richiedono un'adozione mirata, cioè nominativa per casi particolari, causando spesso un irrigidimento da parte delle autorità bielorusse.

Maria, orfana, dieci anni (dovrei dire: signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, ma penso di perdere troppo tempo), provenienza Bielorussia, ospite dei genitori affidatari Chiara e Alessandro Giusto, tenta il suicidio per il terrore di essere rimpatriata, perché ha subìto violenze da parte di ragazzi dell'orfanotrofio, dove, la notte, non esistono controlli. Sarebbe stata più volte spogliata, legata a una sedia o a un letto, costretta a rapporti sessuali con uso di accendini e sigarette. Fantasie di bimba? quanto detto viene certificato da medici della ASL e dall'ospedale Gaslini: «presunta sodomizzazione e segni di bruciature all'inguine.» I genitori, per salvare Maria, la nascondono. Ma Maria non è stata ma rimpatriata. Ieri, una sentenza della Cassazione che dice che i criminali bielorussi presenti in Italia non possono essere spediti in patria perché rischierebbero la vita. Come la mettiamo con Maria, dieci anni, orfana, violentata, che non ha protezione dallo Stato italiano in quanto "non criminale"? Il nostro Stato ha violato la legge e le convenzioni internazionali, facendo prevalere la ragion di Stato. Chiedo al signor Ministro spiegazioni in merito al comportamento della magistratura e del Governo. Troppe sono le connivenze e i misteri che circondano questa disumana storia.

Noi non stiamo parlando della famiglia che l'aveva in affidamento e del suo comportamento, che possiamo giudicare diversamente. Noi stiamo parlando di una notizia di reato che che è stata data con chiarezza, dimostrata dai medici, esplicitata dalle psicologhe e che è stata ignorata. Nella sentenza della corte d'appello di Genova si leggono due cose raccapriccianti: la prima è che non si è ritenuto di sentire la bambina

La prima questione riguarda il nodo dell'adozione. A noi risulta che la famiglia Giusto non ha mai fatto richiesta di adozione della minore in questione; da informazioni assunte dalla Commissione per le adozioni internazionali, risulta che la famiglia in questione ha ottenuto, con decreto del tribunale per i minorenni del 2004, l'idoneità all'adozione per due minori che non sono Maria. Successivamente, nell'anno 2005, la famiglia ha conferito incarico ad un'associazione autorizzata dalla Commissione per le adozioni internazionali per l'adozione di un bambino bielorusso che non è Maria medesima. Tale pratica, però, non è mai stata depositata, essendo stata presentata successivamente al 31 ottobre 2004, data di blocco delle adozioni in Bielorussia. Infatti, le autorità bielorusse non hanno mai accettato il deposito della predetta pratica, adducendo che nuove presentazioni di domande di adozioni avrebbero potute essere effettuate solo dopo il disbrigo delle pratiche di adozione già presenti prima del blocco delle adozioni e ancora attualmente giacenti.

il Governo sia rappresentato dal Ministro nel cui ambito ricade la Commissione che si occupa di questo caso.

ho evitato di commentare la vicenda in ogni singolo passaggio, perché qualsiasi commento che veniva fatto era un ulteriore elemento che rendeva più complicato il difficile lavoro di mettere insieme i diritti della bambina,

dopo che il tribunale dei minorenni di Genova aveva affidato la minore al Comune di Cogoleto per gli accertamenti sanitari, il tribunale stesso aveva disposto il rientro in patria della bambina e si era trovato un accordo in base al quale, nell'ambito di un programma di riabilitazione, la bambina potesse tornare in patria accompagnata sia da un supporto medico e psicologico sia dalla famiglia ospitante.

perché si avevano le garanzie che la bambina non tornasse nella condizione che aveva determinato la violenza, ma si potesse determinare un percorso di reinserimento sociale nel suo Paese di origine,

la bambina non era in Italia per un'adozione, ma per un programma specifico. Noi non potevamo trasformare quel programma specifico in un'adozione; la cosa che potevamo fare era seguire il rientro della bambina per evitare che la stessa si ritrovasse nella condizione in cui si erano determinate le violenze. Ciò è stato fatto,

a costruire un rapporto migliore con la Bielorussia dal punto di vista della verifica delle condizioni effettive in cui i bambini versano negli istituti bielorussi, perché si operava in un ambito

L'ultimo nodo riguarda i problemi relativi ai controlli e al da farsi per evitare che si ripetano casi di questo tipo.

famiglie e associazioni di famiglie - qui parliamo in realtà di associazioni di famiglie - sono in grado di fornire.

negli anni presso la stessa famiglia. Sono tutti nodi che bisogna approfondire. Ripeto, le modalità di verifica delle famiglie, le caratteristiche che devono avere, la ripetibilità dell'affidamento temporaneo, la verifica dei percorsi di formazione, oltre alla sovrapposizione tra richiesta di adozione e pratica dell'affidamento sono tutti nodi che ho chiesto si passassero al vaglio.

affermazione secondo cui, se è successo questo fatto che ha coinvolto una bambina, vuol dire che le nostre procedure non funzionano fino in fondo e sono inadeguate. Avvertire questo da parte del Governo e lanciare anche una disponibilità di collaborazione - come lei ha fatto - verso il Parlamento nel momento in cui, dopo la raccolta del materiale, saranno predisposte le nuove linee guida, credo sia il tentativo

di non chiudere i rapporti con alcuni Paesi perché lasciare uno spiraglio di collaborazione con loro significa anche lasciare aperte le porte della speranza

Nel momento in cui ci si occupa di diritti umani dei bambini e di opportunità da offrire ai bambini, credo che rifarsi alla sola legge, alla sola interpretazione, ferma ed autorevole, del dettato legislativo

e mi verrebbe da dire veramente: «*Sutor, ne ultra crepidam*!» in quanto io, di questo argomento, come Presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia nella precedente legislatura mi sono occupata lungamente e in modo particolare di questi casi, non di una Maria, ma di 30, 40, 50.000 Marie.

CAI, la Commissione per le adozioni internazionali che però, per alcuni aspetti, interviene anche sugli affidi internazionali, e quindi su una materia *in fieri*.

Capisco che lei non ha nemmeno nascosto, signor Ministro, l'imbarazzo di dover rispondere nello stile del *question* *time* inglese che, conosciuto perfettamente solo dal nostro amico Furio Colombo, si presta a risposte "sì o no".

fatto la famiglia Giusto domanda di adozione? Se non l'aveva fatta prima del 13 luglio 2006, risulta comunicato al signor questore di Genova che è stata fatta questa domanda. Precisamente, risulta da un documento, che è in allegato, quanto segue: «in merito alla relazione redatta dal sottoscritto in data 13 luglio, la famiglia Giusto mi ha comunicato che l'associazione alla quale si sono rivolti per richiedere l'adozione avrebbe ipotizzato quale soluzione per la situazione della minore la possibilità di un cambio di istituto». Si era addirittura parlato di cambi di istituto, quindi la domanda di adozione evidentemente c'era. non ha pertanto risposto a questa domanda, così come non ha risposto alla domanda sul perché da dieci anni spesso viene inviato lo stesso fanciullo, la stessa fanciulla, nel posto iniziale visto che, come ho spiegato prima sulla base di una considerazione fatta dall'ENEA - non da me, che sono ignorante in questa materia - bastano due o tre soggiorni. Questo forse allora giustifica - non l'avrei voluto citare, perché sembra quasi che, scritto da questo giornale, si tratti di una qualche speculazione di carattere politico - che in Italia e in Bielorussia ci sia un'industria dei bimbi di Chernobyl perché, sempre che ci si possa avviare verso questa ipotesi di industria, in Italia ben 55 organismi che si occupano di adozione dopo Chernobyl, mentre ce ne sono 10 in Canada e 25 negli Stati uniti. caso riferendomi all'esperienza geopolitica che ha il senatore Colombo, che si tratta di Paesi piuttosto ricchi e, soprattutto, dieci volte superiori per popolazione, per vastità di territorio e per possibilità economiche.

facoltà. VALPIANA *(RC-SE)*. Voglio anzitutto ringraziare il Ministro per il comportamento sottotraccia tenuto in tutta questa vicenda e per la sobrietà con cui anche oggi ha affrontato questo caso. Sobrietà della quale ci sarebbe stato sicuramente bisogno in tutta questa vicenda di Maria, ma, io credo, in tutta la partita

con la Bielorussia, che, ricordo, è uno Stato sovrano. Di tanti bambini si abusa in Italia, in Francia, in Belgio, ma nessuno si è sognato di mettere in discussione la capacità di questi Stati di fare giustizia e di rendere giustizia a questi bambini colpendo i colpevoli. Non capisco perché con la Bielorussia ciò sia stato fatto,

Maria, in tutti i tanti casi di bambini italiani e stranieri come quello di Maria, potrebbe essere una figura importante che tutela il diritto soggettivo di ogni bambino, visto - speriamo - non come

in Aula confondendo affido, soggiorni e adozione) di grandi campagne di informazione per chiarire a tutti i cittadini italiani la differenza tra questi istituti giuridici.

il caso di Maria impone un'importante riflessione, che abbraccia tutti i bambini bielorussi e le innumerevoli coppie italiane che soffrono da anni per coronare il loro desiderio di adozione. Queste famiglie desiderano dare amore, ma si trovano costrette, a causa di un meccanismo perverso, a pagare denaro per potere dare questo amore. È incredibile! Ancor peggio, si tratta di famiglie "interrotte": tre mesi d'estate e poi un lungo inverno, fatto di voli aerei, regali, sofferenze, disagi, alberghi e impegno economico per sostenere gli istituti che ospitano i bambini (medicinali, servizi igienici minimi, aule scolastiche). Ci credo che occorra tanto tempo per riuscire a ottenere l'adozione di un bimbo bielorusso! I viaggi tra genitori e bambini coinvolti nel programma rendono tra i 132.000 e i 136.000 euro l'anno, cifre tali che - come sostiene il Ministro - vengono tenute in conto nella finanziaria bielorussa. I bambini in affido sono, di fatto, un*business*

dell'amnesia. Ritengo necessario andare in Bielorussia, dove Dario e io siamo molto conosciuti perché da oltre dieci anni vengono rappresentate le nostre commedie: in questo momento, proprio a Minsk, è in scena

spero sia vero - gli orfanotrofi in Italia entro dicembre. Me lo auguro veramente e spero anche che le pratiche per le adozioni vengano sveltite e che tanti bambini senza sorrisi possano trovare finalmente l'amore e il calore di una famiglia, di una madre e di un padre.

Signor Ministro, vorrei dirle grazie anch'io, come hanno fatto i colleghi, perché certamente ha aggiunto molte cose importanti. Tuttavia, ha scelto - lo noto con dispiacere - di non rispondere a nulla

Una sola bambina risulta essere stata oggetto di violenze inaudite. Tali violenze sono state fisicamente accertate da medici pubblici delle ASL e non da strutture private. Sono state psicologicamente accertate da esperti che hanno scritto per i due tribunali (tribunale e corte d'appello) cose drammatiche e sono avvenute in Bielorussia. Signor Ministro, se si tratta di un adulto del cui comportamento immorale in Thailandia giunge notizia a Milano, la giustizia interviene a Milano e non lo rimanda certo in Thailandia.

Ho cercato di avere rapporti con i migliori «cervelli» italiani in materia di psicologia infantile: la riabilitazione mentale non esiste. é un processo di presa di possesso da parte di uno Stato. È stato detto che nessuno deve essere proprietario, lo ha detto la senatrice Valpiana facendo uno sprezzante riferimento ai coniugi Giusto, che hanno avuto la terribile colpa di volere bene

con riferimento all'atto ispettivo cui si risponde, relativo ai lavori di realizzazione della terza corsia sulla A9 nel tratto Como Grandate - Lainate, si fa presente che, in data 15 giugno 2006, la commissione per la VIA ha espresso il parere di compatibilità ambientale per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A9 nel tratto Lainate-Como. Il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare, per quanto di propria competenza, fa conoscere che nel corso della valutazione tecnica effettuata da parte della predetta Commissione sono emersi alcuni significativi elementi di criticità. Questi hanno riguardato, in particolare, l'impatto provocato dall'inquinamento atmosferico ed acustico sui territori coinvolti fortemente antropizzati e che presentano particolari rilevanze ambientali. Tali elementi hanno determinato, pertanto, l'emanazione nello stesso parere della Commissione di alcune prescrizioni volte proprio a superare dette criticità. Attualmente, la commissione per la VIA sta procedendo ad una circostanziata disamina della questione inerente le problematiche emerse al fine dell'emissione del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale. Nelle more del suddetto pronunciamento, la Conferenza di servizi, tenutasi da ultimo lo scorso mese di agosto, non può essere chiusa. Per quanto attiene, infine, le previsioni di conclusione dei lavori, va segnalato che, così come indicato nel piano finanziario allegato al IV atto aggiuntivo sottoscritto tra ANAS ed Autostrade per l'Italia S.p.A., una volta conclusa la conferenza dei servizi occorreranno circa tre anni per arrivare al completamento dell'opera.

Signor Presidente, desidero ringraziare il sottosegretario Casillo per la consueta cortesia con cui risponde ai numerosi atti di sindacato ispettivo che, anche con altri colleghi

nel merito queste criticità perché, dal nostro punto di vista, quando si parla di inquinamento ambientale, nulla può essere peggiore di quello che

che, parlando a proposito di Pedemontana, di Brebeni e di terza corsia, ha agghiacciato gli operatori economici lombardi e anche i rappresentanti del Parlamento. Abbiamo la sensazione che il ministro Pecoraro Scanio abbia intenzione di fare della terza corsia quanto è stato fatto, ad esempio, della Pedemontana, cioè un progetto atteso per circa 40 anni. Ora non è più possibile attendere. Ringrazio il sottosegretario Casillo,

Per quanto concerne i tempi, sottolineo che allegato ad un settimanale (ora non ricordo se fosse il *Magazine* del «Corriere della Sera») vi era un opuscolo, patrocinato anche dal Ministero, che spiegava chiaramente come entro il gennaio 2009 quell'arteria sarebbe stata pronta.

da rivendicare. È assolutamente necessario ed urgente per l'economia lombarda che si realizzi la terza corsia e si razionalizzi lo svincolo fra l'A9 e l'A8.

n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, ha differito al 31 dicembre 2006 il termine previsto per l'emanazione del decreto interministeriale per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi, al fine di consentire il razionale completamento degli accertamenti tecnici relativi alle attività connesse alla revisione dei canoni stessi. Nel contempo, il disegno di legge finanziaria per il 2007, attualmente all'esame del Parlamento, reca all'articolo 16 una disposizione che detta nuovi criteri di quantificazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime, nell'ottica di perseguire obiettivi di equità e razionalità. Ricordo agli onorevoli senatori che vi era stata nella passata legislatura una norma introdotta da una legge finanziaria con la quale si aumentava il canone delle delle concessioni marittime di ben il 300 per cento. Vi sono state, proprio su sollecitazioni delle Regioni, svariate proroghe, l'ultima delle quali fu chiesta proprio dal Ministro del turismo,

nella legge finanziaria sia improntata a criteri di equità e razionalità.

nell'articolo 16 della finanziaria che la Camera sta esaminando. Quindi, da questo punto di vista bene facemmo a raccogliere quell'invito delle Regioni e delle categorie

della lotta all'abusivismo e che quindi, attraverso il tavolo tecnico e il rapporto tra Regioni e categorie, andava affrontato proprio il tema della classificazione, differenziando le varie aree - in un Paese come il nostro non c'è dubbio che le aree sono diverse - ed emanando norme chiare. Ringrazio

dell'iniziativa delle Regioni. Rispetto alla proposta contenuta in finanziaria mi sembra che le due priorità da lei richiamate, equità-razionalità e superamento, finalmente, di un regime di incertezza per gli operatori (perché quei rinvii, seppure evitavano gli aumenti, determinavano incertezza), siano già sufficienti. I tre assi che ho colto nella finanziaria sono: la classificazione legata alla qualità,

che ritenevamo iniqui e indiscriminati gli aumenti precedenti: iniqui, perché non assumevano il carattere produttivo delle aree demaniali, soprattutto quelle legate alla balneazione (oggi questo ruolo produttivo viene colto dalla finanziaria, anche con le differenziazioni previste);

il concetto dell'obbligo di transito. Esso va distinto, a mio avviso, fra concessioni esclusive e non esclusive, sia per salvaguardare la sicurezza dei bagnanti, la tutela della loro salute e dell'ambiente, sia per favorire l'aumento delle entrate, perché la concessione esclusiva prevede un canone doppio.